una nuova finestra"). Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

Pertanto, procediamo con l'esame degli emendamenti sui quali l'*iter* della Commissione bilancio si è concluso. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 01.1, 3.10, 3.102 (già 3.15), 3.35 (testo 2), 3.105 (già 3.49), 4.0.1 e 5.0.15. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 5.0.100.

Grazie che sancisce anche oggettivamente il fallimento del provvedimento sulle liste d'attesa. Abbiamo assistito a un conflitto istituzionale senza precedenti tra la Conferenza Stato-Regioni e il Governo, che ha portato di fatto a uno svuotamento del cuore di un provvedimento che, d'altra parte, è nato senza un sostanziale apporto finanziario che permettesse anche soltanto di attuare le misure che il provvedimento con sette decreti attuativi previsti che vanno alle calende greche, tre dei quali addirittura senza neanche una data di scadenza. Quindi, di fatto, questo provvedimento purtroppo avrà un esito solo, cioè che per i cittadini italiani non cambierà niente. Sull'articolo 2, in particolare, la mediazione (se così si può chiamare) uscita fuori dalla Commissione su proposta del Governo di fatto crea soltanto un nuovo organismo burocratico all'interno del Ministero della salute, per cui si farà un nuovo dirigente e verranno assunte nuove persone, che di di fatto va a sovrapporsi a organismi già esistenti, che potevano essere rafforzati e utilizzati per il raggiungimento del monitoraggio dei dati e del funzionamento delle attività delle Regioni. Soprattutto, all'articolo 2 si sancisce politicamente che ci sono due anime in questo Governo: una che procede, da un lato, sull'autonomia differenziata (d'altra parte, votata dalla maggioranza) e l'altra che invece lavora sull'accentramento delle funzioni a livello statale, costruendo una contrapposizione istituzionale e costituzionale che che pagano i cittadini, perché, a quasi due anni dall'inizio di questa legislatura, non abbiamo ancora sul tavolo una riforma della sanità che risponda ai bisogni del Paese dopo il Covid *(Applausi);* non abbiamo una riforma sul personale sanitario; non abbiamo una riforma sui salari del personale sanitario; non abbiamo una riforma sui tempi di lavoro; non abbiamo una riforma sulle specializzazioni e ci troviamo ancora una volta con gli *slogan* della campagna elettorale, che però è finita e quello che rimane è un provvedimento vuoto.

Signora Presidente, mi auguro di ricevere aperture da parte della maggioranza rispetto agli emendamenti che ho presentato all'articolo

costi aggiuntivi, ma che porterebbe solo miglioramenti nella vita dei pazienti affetti da patologie oncologiche, che si ritrovano (come sempre, purtroppo, per quanto riguarda la sanità), a vedere azioni a macchia di leopardo e diversificate da una Regione all'altra con notevole aggravio per loro e i loro *caregiver* per quanto attiene alla prenotazione di esami, visite, controlli, terapie e chi più ne ha più ne metta. Con linee guida chiare da parte del Ministero potremmo quindi agevolare la

perché prevede che nel momento in cui un cittadino presenta una richiesta di prestazione a un'azienda sanitaria, sia questa a farsi carico dell'onere di trovare un appuntamento, nel rispetto delle tempistiche del codice di priorità stabilito dalla prescrizione medica, che è quanto di più logico. *(Brusio).* PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché è davvero complicato ascoltare chi parla. PIRRO Ciò è quanto di più logico possa accadere, laddove l'azienda è obbligata per legge al rispetto delle tempistiche. Bastava questa semplicissima norma a risolvere i problemi dei cittadini

che deve garantire il direttore di un'azienda sanitaria non sono infatti tanto di natura economica quanto in termini di prestazioni erogate ai cittadini e allora c'è di più semplice che prevedere che, laddove non raggiungano il risultato di ridurre le liste d'attesa o di esiti di salute dei cittadini assistiti dalle proprie aziende, abbiano non un 30 per cento di riduzione di questa retribuzione di risultato? Mi sembrano norme di tale buon senso che mi auguro di vedere uno spiraglio nel relatore e nel Governo in merito all'accoglimento di queste proposte, a mio avviso così sensate e utili ai cittadini italiani, di cui tutti ci dovremmo preoccupare, ma di cui forse non ci preoccupiamo abbastanza.

durante le audizioni. Vorrei evidenziare come non solo questo Governo non abbia ascoltato e non abbia recepito praticamente nulla

Tale emendamento è stato suggerito durante le audizioni e, come dicevo, il Governo non ha ascoltato neppure i pareri di chi è venuto in audizione a manifestare qualche perplessità. perplessità. Si tratta, tra l'altro, di un emendamento a costo zero. Capisco che siano state bocciate proposte che prevedevano una spesa, ma per gli emendamenti a costo zero come questo davvero mi chiedo il Qui si dice che per rinnovare l'accreditamento del privato che opera in ambito sanitario bisogna prevedere un prerequisito, e cioè che quel privato abbia rinnovato i contratti del personale sanitario. Ci sono strutture private che lavorano con personale che ha un contratto scaduto vent'anni fa. Cosa costava dire che per accreditare il privato serve quantomeno che esso paghi in maniera dignitosa il personale sanitario? Non venite a raccontarci che per voi il personale sanitario è una priorità. Se non prevedete nemmeno che per accreditare il privato serva rinnovare contratti scaduti vent'anni fa, mi chiedo in che modo intendiate valorizzare il personale sanitario.

Unit, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas che hanno una struttura organizzativa multidisciplinare. Faccio notare a tutti che dalle ultime statistiche a livello europeo quello del pancreas è il tumore che sta avendo la maggiore diffusione su tutto il territorio europeo, probabilmente anche condizionato dai nostri stili di vita. In ogni caso, questo tipo di tumore ha bisogno di una particolare cura, soprattutto a livello chirurgico. In Italia ci sono centri per le Pancreas Unit, ma non sono diffusi su tutto il territorio.

che con noi ha realizzato un percorso per cercare di sollecitare Agenas alla realizzazione di linee guida per le Pancreas Unit. Ci tengo quindi a sottolineare la sensibilità di tutti e, quando voteremo, spero che tutti i senatori e tutte le senatrici possano aggiungere la firma a quest'ordine del giorno.

in cure primarie e territoriali che sono gli unici specialisti non in grado di operare in tutti gli ambiti in cui si formano.

hanno stabilito gli ambiti formativi e hanno statuito che questi specialisti in cure primarie si formano anche per operare nell'ambito della medicina generale, seguendo tra l'altro *standard* formativi europei. Ebbene, poiché c'è un potente sindacato di medicina generale che evidentemente si oppone a che questi specialisti possano operare nell'ambito della medicina generale, noi stiamo impedendo a medici già formati di essere impiegati

davvero che i pareri del relatore e del Governo siano favorevoli a questo emendamento, che è assolutamente necessario, perché qui abbiamo professionisti che stanno subendo da vent'anni una mortificazione che impedisce loro di lavorare nell'ambito in cui si sono formati.

perché in Conferenza Stato-Regioni il Governo si era reso disponibile a modificare il comma 2 dell'articolo 5, che prevede le 5, che prevede le modalità per determinare il fabbisogno di personale sanitario nelle singole Regioni. Nel decreto-legge è riportato che lo si fa attraverso un decreto

non è finita qua. Dopo aver approvato il fabbisogno di personale, si deve emanare un altro decreto per autorizzare la spesa. A me sembra che la volontà del Governo di abbattere effettivamente il tetto di spesa per il personale sanitario sia fittizia e lo dimostra proprio questa cosa. Oltretutto, noi siamo stati bloccati in Commissione per giorni e giorni proprio su questa diatriba fra Regioni e Governo. L'articolo 2 è stato modificato. Aspettavamo anche la modifica dell'articolo 5 proprio su questo punto, modifica che non è arrivata. Per questo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo di questo ultimo pezzo del comma 2, perché

G5.100, la *ratio* è sempre quella di reperire personale sanitario, soprattutto medico, già disponibile da utilizzare per accorciare le liste d'attesa, su due ambiti. Abbiamo presentato emendamenti in materia, ma anche un ordine del giorno che sostanzialmente dice la stessa cosa, ossia propone di eliminare il vincolo che oggi impedisce ai medici in formazione specialistica di esercitare anche la libera professione intramuraria negli ospedali. se noi togliessimo quel vincolo - quantomeno, per esempio, per i medici specializzandi al quarto o quinto anno - potremmo avere personale disponibile per accorciare le liste d'attesa. I medici lo chiedono da moltissimo tempo. Tra l'altro, ci chiedono giustamente anche di trasformare il loro contratto, che è di formazione, in uno di formazione-lavoro, visto che questi medici in formazione fanno turni veri e propri e quella non è formazione, ma lavoro. Mi rendo conto che per trasformare un contratto di formazione

si occupa di un settore che voi continuate a dimenticare, quello dell'emergenza-urgenza territoriale (il 118 e le ambulanze). Questi sono gli unici operatori sanitari per i quali non è previsto nessun riconoscimento del rischio biologico biologico e lavorativo. Eppure il personale che lavora nell'emergenza-urgenza territoriale, sulle ambulanze, è esposto ad altissimi rischi. Questi sono gli operatori che ci aiutano a gestire le emergenze, i terremoti o le alluvioni. Ma com'è possibile che per questi medici, che operano in altissime condizioni di rischio, per questi infermieri e per questi volontari non siano riconosciuti il rischio biologico e il rischio ambientale?

Signora Presidente, uno dei pochi aspetti positivi, se vogliamo trovare qualcosa di positivo in questo decreto-legge, è che quantomeno ci sia un articolo dedicato alla salute mentale, spesso ultima cenerentola della sanità, con tantissimi problemi, questioni e nodi da risolvere. Una delle cose più sentite da chi si occupa del tema e da chi tutti i giorni passa la vita a gestire persone affette da problemi di salute mentale è avere a disposizione dei centri polifunzionali che possano prendere in carico e occuparsi delle persone con questo genere di difficoltà a 360 gradi, in una maniera appunto multidisciplinare, che è un termine che usiamo sempre di più quando parliamo di salute e sanità. La richiesta che arriva da tutte le associazioni, da tutti i pazienti, è di avere la possibilità di un approccio multidisciplinare. Ciò è ancor più valido quando si tratta di persone con problemi di natura mentale. Allora, bastava poco per dare un segnale vero a chi ha tanti problemi relativi a questa sfera: accettare un emendamento di indirizzo, perché di ciò si tratta in questo articolo, semplicemente di linee di indirizzo. Eppure, anche su cose di buonsenso come questa, in Commissione, è stato dato parere contrario. Io mi auguro auguro che, arrivato all'attenzione di quest'Assemblea, il tema possa avere la dignità e il rispetto che merita e l'attenzione da parte di tutti noi.

avanzata per il trattamento dei tumori, cioè la protonterapia per tumori localizzati in aree critiche e difficilmente raggiungibili con le tecniche tradizionali di radioterapia.

tra le Regioni affinché nel Sud Italia vi sia un trasferimento di conoscenze e tecnologie su questa importante modalità di trattamento dei tumori.

uno strumento per risolvere il problema delle liste d'attesa, non si capisce perché questo emendamento, come anche altri simili, non vengano presi in considerazione, dal momento che essi vanno semplicemente ad evitare che si perda il beneficio del taglio del cuneo fiscale introdotto nell'ultima legge di bilancio, con il superamento della soglia dei 2.600 euro. Chiedo appunto alla maggioranza di riflettere nuovamente su questo punto. C'è molto personale coinvolto da questa penalizzazione e, quindi, credo che faremo un favore a tutti.

esprimo parere favorevole con riformulazione dell'impegno in: «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di

«a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di

che esso venga preso in considerazione dal Governo perché potrebbe dare una grossa mano per risolvere il problema della carenza infermieristica e per omogeneizzare le mansioni all'interno dei reparti.

l'opportunità di». Questi due ordini del giorno affrontano due argomenti molto importanti. Il primo chiede di poter utilizzare personale medico già disponibile, e in particolare i medici specialisti,

C'è sempre stata un'apertura anche da parte dello stesso Ministro verso questo tema e, quindi, almeno valutiamo l'opportunità di lavorarci in futuro. Il secondo ordine del giorno, G 5.100, chiede invece di immaginare di immaginare per i medici e per gli operatori che operano nell'ambito della urgenza territoriale che vengano valorizzati non solo come figura professionale - oggi sono gli unici per i quali non è previsto

Signor Presidente, pochi temi come la sanità minano in profondità la fiducia fra lo Stato e i cittadini e pochi temi, come le interminabili liste d'attesa, suscitano indignazione e rabbia. Pensiamo tutti che sia inaccettabile il trascorrere di mesi, qualche volta di anni, prima di poter fare una TAC o una mammografia. ovviamente, come ci ricordano i medici, ha un effetto economico e anche sul tema della prevenzione e sulla salute dei cittadini. È quindi evidente che il diritto alla salute rappresenta la prima preoccupazione dei cittadini. Di fronte ai cambiamenti strutturali, come l'invecchiamento della popolazione e i ritardi interminabili dopo il Covid-19, tutto questo porta alla necessità e all'urgenza di una riorganizzazione della sanità. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e, poiché siamo intellettualmente onesti, non attribuiamo la responsabilità di questa vera e propria emergenza solo a questo Governo e, anche dai banchi dell'opposizione, proviamo a fare la nostra parte. Come ha ricordato recentemente la Corte dei Conti, la spesa sanitaria *pro capite* è la metà di quella tedesca e purtroppo la previsione per i prossimi anni parla di un definanziamento della sanità, così com'è evidente a tutti la scarsità di risorse umane: è diminuito di 25.000 unità il servizio sanitario nazionale. Questi dati, con questa scarsità di risorse economiche ed umane, e la sfida

è pregato di allontanarsi; diversamente, di abbassare il volume e consentire a tutti noi di seguire il dibattito in Aula. a questo quadro, credo che la politica sia chiamata ad evitare contrapposizioni sterili e a mettere davvero da parte ogni forma di partigianeria e di ideologia per provare a trovare delle soluzioni. D'altronde, il nostro non è l'unico Paese alle prese con questa sfida: è toccato in Gran Bretagna al Governo di Tony Blair, che ha dovuto affrontare una riforma della sanità e lo ha fatto sicuramente stanziando più risorse, ma al tempo stesso puntando sull'integrazione dei servizi, su una maggiore formazione da parte degli operatori sanitari, sulla valutazione delle *performance* e anche sul maggior coinvolgimento dei privati. Purtroppo in Italia le cose stanno andando diversamente. Abbiamo assistito a una tensione con le Regioni, anche con quelle che hanno lo stesso colore politico maggioranza. Il principio ispiratore di questo provvedimento lo ha ricordato ieri Carlo Calenda e noi lo condividiamo. La volontà di abbattere le liste d'attesa è ovviamente un fatto sacrosanto, però è chiaro che il decreto-legge in esame mette in ordine alcuni interventi che sarebbero anche di buon senso; lo ha sottolineato durante le audizioni Walter Ricciardi, che ha giustamente ricordato come non basti l'aumento delle risorse, ma serva incrementare il personale, migliorare la gestione, puntare sulla telemedicina, sulle cartelle cliniche elettroniche e anche - perché no - sull'intelligenza artificiale e su un maggior coordinamento tra gli ospedali e il territorio. Queste misure quindi non solo da noi sono condivise, ma durante l'*iter* della precedente legge di bilancio, come Azione, avevamo avanzato esattamente le stesse proposte. Cosa non ci convince e cosa non funziona all'interno del provvedimento? Sappiamo tutti che per abbattere le liste d'attesa servono almeno due miliardi, in un contesto nel quale è ormai quasi certo il ritorno dei vincoli rigidi del Patto di stabilità. Se questo decreto-legge è stata la risposta del Governo e della maggioranza, è chiaro che stanziare un quarto delle risorse necessarie per abbattere le liste d'attesa non è quello che ci saremmo aspettati. Consentitemi però di dire che la retorica opposta, quella utilizzata dall'opposizione e dal Partito Democratico, non ci convince. L'abbiamo fatto tutti, ma qualche volta credo che su un tema così serio come questo si debba evitare dell'opposizione coperture che di fatto sono sostanzialmente molto difficili, se non impossibili. Noi pensiamo che, tra la scarsità delle risorse stanziate dalla maggioranza e la moltiplicazione dei pani e dei pesci da parte dell'opposizione, quest'Assemblea dovrebbe fare un supplemento di riflessione e anche con dei sacrifici, perché è chiaro che trovare queste risorse non è facile. Se però pensiamo davvero che quello alla salute sia il primo diritto che la Carta costituzionale garantisce, qualcosa in più bisogna fare e questo provvedimento sicuramente non basta. Siamo quindi chiamati tutti a trovare delle risorse; noi come Azione lo abbiamo fatto, pescando anche da un provvedimento provvedimento doloroso, perché il taglio al cuneo fiscale per noi è una cosa seria. Se però le risorse non ci sono, due miliardi si possono prendere anche dal taglio del cuneo pur di evitare e di contrastare le liste d'attesa. Se poi ci sono risorse che avanzano sul reddito di cittadinanza, utilizziamo quelle prima di incidere sul taglio del cuneo, ma utilizziamo coperture vere diamo ai cittadini risorse vere per abbattere le liste d'attesa. Noi purtroppo pensiamo che questo provvedimento, che nelle linee di indirizzo sarebbe pure simile alle proposte di Azione, non raggiunga il risultato,

Signora Presidente, colleghi e colleghe, membri carissimi del Governo,

che hanno vissuto con me per tanti anni - a proposito, auguri al presidente La Russa La Russa - mi permettono, con l'umiltà che non ho sentito mai ieri dai membri dell'opposizione, di fare alcune considerazioni che arrivano ad oggi. Ho sentito dire oggi che la Germania complessivamente spende più di noi. Non è questo che conta, quello che conta è spendere bene. In Germania credo che esistano ancora i manicomi manicomi e non esiste una reale integrazione scolastica. Perché ne parlo? Perché io, pur essendo belloccio, bravino e ora pure abbronzato, riuscivo a camminare dopo tanti anni, ma sono stato rifiutato a scuola fino al liceo e sono riuscito a vivere a spese dei miei parenti. Mia mamma, Leonilde, una grande leonessa,

perché mentre stavo lì a patire la solitudine, sentivo per strada, nel quartiere Flaminio, sciamare i miei colleghi, piccoli alunni, ridere, scherzare, fare le botte e imparare il gioco meravigliosamente crudele della vita. A me quel cavolo di banco azzurro mi è rimasto impresso, lo ricordo tutte le sere. Poi ho avuto qualche piccolo successo e qualche piccolo momento di vita vera, anche oggi, ma le ferite create da quel banco fasullo non me le ha mai levate nessuno, nemmeno oggi che ho il grande onore di parlare come membro del Senato in quest'Aula, perché certe realtà che ti si negano ti rimangono per sempre. Allora io sono orgoglioso di questo Paese che combatte contro il sorvegliare e il punire e che cerca di sostenere la scuola di tutti per tutti, perché, se cominciamo

un attacco totale della minoranza a qualcuno di noi definendoci brutti, sporchi e cattivi, ma dando l'ho seguito con attenzione, anche se nel rispetto delle minoranze, con un po' di preoccupazione e di ribrezzo

- a tre emendamenti della maggioranza per migliorare la possibilità di donare il sangue attraverso più che il politico, in questo caso. Oggi è andata un pochino meglio, c'è un clima leggermente più positivo. Perché dico questo? Perché non si può delegittimare senza proporre, dicendo che questo provvedimento è uno *spot* elettorale: a parte che non è vero, ma si vota talmente spesso che qualsiasi provvedimento purtroppo diventa, per coincidenza anche non voluta, uno *spot* elettorale. Vogliamo cominciare a entrare nel merito, colleghi? *(Applausi)*. Proponiamo cose alternative. Io faccio il medico, posso criticare il collega per una terapia, persino la psicoterapia la considero in certi casi, pur praticandola, un momento di oppressione invece che di liberazione, a seconda di chi la fa. Ho un po' la puzza sotto il naso e mi sono fatto qualche avversario, ma mai nemico. Forse è questo quello che ieri mi è venuto in mente con più forza. Ma perché, se si pensa in maniera diversa - mi viene il dubbio che non si pensi affatto, ma lasciamo stare l'avversario deve diventare un nemico da delegittimare ad ogni costo? Persino il mio scooterino tanto carino può diventare un momento di oppressione per chi non sa capire quanto mi costa non usare più le mie gambe

quasi tutto quello che è in corso di discussione appartiene all'apparato regionale

se il Governo Meloni, che condivido con il cuore, si è preso l'impegno di ridiscutere riproporre in maniera realistica e concreta, certo sapendo benissimo la complicatezza di quello che si vuole discutere, chi ce l'ha fatto fare? Ce l'ha fatto fare il voler riproporre con forza, anche con dolore, un argomento essenziale, perché - e lo dice uno che non si è negato qualche malattia, oltre alla cura degli altri - l'attesa è qualcosa di incredibilmente negativo. Questo non lo dicono solo le associazioni che stimo, ma anche io stesso.

perché dobbiamo riproporre con coraggio e non con delegittimazione sciocca l'argomento dell'attesa, perché ripropone l'intero assetto della sanità, della salute e della prevenzione in questo periodo post-pandemico su cui

ogni volta che parlo in quest'Aula *(Applausi),* perché credo che qualcuno mi ascolti; magari mi delegittima, ma è sempre un momento di storia,

persone che non conoscerò mai, forse quelle che contano di più: non ti conoscono, non ti votano e non ti dovranno mai dire grazie (perché anche dire grazie è un ricatto). Ma io oggi mi sento libero di parlare con voi, sapendo che qualcuno mi apprezzerà; tanti mi dimostreranno dimostreranno di essere contrari e li ringrazio, perché essere contro un disabile è sempre un momento di parificazione senza pietismo (quello che non ha Maria Giovanna quando è dura con me: insomma, mi picchia e cerco di evitarlo, perché è più alta di me e più forte). Signora Presidente, ogni mattina il gallo canta, fa chicchirichì e dice: vedi quanto sono potente? Il sole sorge perché dico chicchirichì. Ragazzi, amici e amiche, non fate chicchirichì. Collaboriamo insieme, anche dimostrando di non apprezzare certi momenti, ma senza deliri di onnipotenza, che fanno male a tutti, e senza - concludo davvero e mi scuso - vedere l'avversario come un nemico, perché io non ci sto: all'avversario che mi dimostra di essere tale io do una carezza, ma se mi vede come un nemico, io gli do un cazzotto e so come farlo. Grazie Presidente e viva la vita. Senatore Guidi, posso rassicurarla sul fatto che la Presidenza è custode del dibattito dell'Assemblea, delle libertà e, ovviamente, anche della vivacità Signor Presidente, quello delle liste d'attesa è uno dei problemi più gravi del nostro sistema sanitario.

se da un lato condividiamo l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa, dall'altro non condividiamo il metodo alla base di questo provvedimento. Serviva un confronto preventivo con le Regioni e le Province autonome. Si è deciso invece di calare dall'alto, nella forma di un decreto-legge, decisioni che poco si conciliano con la natura regionalista del Servizio sanitario e il principio di leale collaborazione che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra lo Stato e le Regioni. In particolare, con l'articolo 2 si stava andando a intaccare una competenza che è in capo alle Regioni, quasi con un paradosso: da un lato l'autonomia differenziata, dall'altro una legge su una materia così sensibile con un deciso profilo centralista. Questo è stato ancora più grave per le Regioni e le Province autonome, le quali - va sottolineato - provvedono autonomamente al finanziamento del sistema sanitario con risorse interamente provenienti dal proprio bilancio. In tal senso, è doveroso ricordare in quest'Aula la sentenza n. 80 del 2007 della Corte costituzionale, la quale indica espressamente che le funzioni di verifica delle liste d'attesa rientrano nella potestà legislativa ed amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione di istituzioni ed enti sanitari, attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il confronto successivo, con l'accoglimento di alcuni nostri emendamenti, è riuscito a mitigare il rischio di una lesione delle prerogative delle autonomie Le nostre competenze vengono salvaguardate, anche se permangono ancora alcune criticità. Per questo motivo, abbiamo ripresentato in Aula emendamenti all'articolo 2 per l'esplicita esclusione delle autonomie speciali e sulla clausola di salvaguardia rinforzata, che purtroppo non sono stati accolti. accolti. Presidente, per affrontare davvero il problema delle liste d'attesa servono risorse e personale; senza di essi il riconoscimento e il rimescolamento della *governance* o l'esercizio di indebite pressioni sulle Regioni sono solo un gioco a somma a somma zero. Nella nostra terra siamo ogni giorno impiegati per garantire una sanità pubblica sempre all'altezza e questo nonostante il problema, ormai cronico, di carenza di personale medico e paramedico. Ringraziamo il relatore, il Presidente della Commissione e il Governo per le migliorie al testo e per il clima di attenzione e ascolto che c'è stato questa settimana in Commissione. Come lei sa, Presidente, nel nostro Gruppo convivono sensibilità e provenienze politiche differenti, pertanto ciascuno di noi esprimerà liberamente il proprio voto sul provvedimento al Signora Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il tema della sanità meritava un dibattito più alto di quello che abbiamo fatto, non tanto noi in Parlamento, in Senato, nelle Commissioni, ma noi come soggetti politici. Ho molta stima del senatore Guidi, che però si è lamentato del fatto che abbiamo definito uno *spot* elettorale un decreto-legge sulle liste d'attesa annunciato ai TG nella settimana precedente alle elezioni europee:

Mi scusi, senatore Renzi, senatore Paroli, rischiamo di sentire più lei che il senatore Renzi. portare alla buona educazione il senatore Lotito è un'operazione alla quale neanche la Presidenza del Senato potrà mai arrivare. Quindi apprezzo il suo tentativo di chiedere a Lotito di essere una persona… PRESIDENTE. Però stavolta è incolpevole. Lotito è quello sopra, quindi tranquilli, non è un problema. È però la dimostrazione, in una foto, di quello che sta facendo questa maggioranza: utilizza il tema della sanità per prendere un voto, ma non affronta le questioni reali, facendolo a a fronte di una disponibilità di tutte le opposizioni, in modo diversificato, a dare davvero una mano su questi temi. Non lo avete fatto, colleghi, e avete scelto la strada della propaganda. Dall'altro lato, signora Presidente, questo atteggiamento populista è confermato da chi dice - in questo caso, dall'opposizione - che negli ultimi vent'anni tutti i Governi hanno tagliato. Siamo in presenza di un dibattito falso, di una *fake news* trasformata in dibattito parlamentare. Non è vero che le liste d'attesa si risolvono con questo decreto-legge e non è vero che negli ultimi vent'anni tutti i Governi hanno tagliato. È vero invece il contrario, che tutti i Governi hanno investito di più, magari non a sufficienza, magari non quanto vi sarebbe stato bisogno, ma tutti i Governi hanno messo più soldi. Solo che, nel dibattito politico, il racconto è sempre lo stesso. Faccio degli esempi concreti. Quando nel 2014-2015 la collega Lorenzin, allora Ministra, mise un miliardo di euro in più sul fondo sanitario, quel miliardo di Sul fondo farmaci innovativi. Sapete cos'è quel fondo farmaci innovativi? È il fondo che finanzia la risoluzione dei problemi - lo

a dire che non si sono messi soldi in più. E sono populisti anche quelli che, dall'opposizione, dicono che tutti i Governi hanno tagliato e adesso arrivano loro. Non è così. Tutti i Governi hanno messo più soldi; il punto è dove sono stati

centralizzazione degli acquisti: è un'operazione lanciata dall'ex collega Gutgeld, allora commissario per la revisione della spesa. Viene lanciata nel 2014 ed entra in vigore nel 2016-2019. Nel 2016-2019 i bandi per l'acquisto

c'è un risparmio del 23 per cento (cioè lo sconto medio sull'acquisto è del 23 per cento). Quando lo faceva il singolo ospedale, lo sconto medio era del 4 Capite cosa significa questo? Significa che ci sono circa 6-7 miliardi di euro all'anno di risparmio per lo Stato, che non è che sono messi in bilancio con un segno negativo davanti sulla sanità, ma vengono spesi per altre questioni. Questo vostro dibattito sul mettere un miliardo in più o un miliardo in meno intanto è falsato, perché basterebbe un qualsiasi normale studente di economia per capire che mettere un miliardo di euro in più quando c'è la deflazione spero di non dover spiegare cosa sia), cioè quando sostanzialmente il costo della vita è piatto, è diverso dal mettere un miliardo in più quando c'è l'inflazione. È vero che in questi anni il Governo ha messo più soldi, ma, se l'inflazione solo per la bolletta energetica dell'ospedale si mangia tutto l'aumento, è chiaro che stiamo prendendo in giro i malati, una volta di più. Ed è inutile che il Governo continui a dire "abbiamo messo più soldi di tutti gli altri", perché per forza ogni anno si mettono più soldi: è un aumento, come dire che quest'anno voi siete i *recordman* del debito pubblico; è ovvio, perché ogni anno si aumenta il debito pubblico, ma questo richiedeva un ragionamento serio e non

le malattie rare hanno totalmente modificato il proprio impatto sulla vita quotidiana. Negli ultimi tre anni l'età media (l'aspettativa di vita) è cresciuta di un anno. La mortalità o, meglio, più correttamente, la riduzione della mortalità per le malattie croniche - è del 35 per cento. Oggi chi ha una diagnosi di tumore vive in media molto più a lungo di quello che accadeva vent'anni fa. Capite che questi argomenti, legati all'allungamento dell'età media, portano a un cambio radicale? Quali sono i nostri punti di forza? La tecnologia, signora Presidente, di cui non si è parlato, se non per *spot*. L'intelligenza artificiale è il nostro alleato più grande nella gestione più grande nella gestione della sanità. Ci sono Paesi - il Sudafrica, l'India o i Paesi asiatici - che stanno investendo nell'intelligenza artificiale per la gestione degli infarti gestione degli infarti e oggi almeno 10 milioni di casi di infarti sono gestiti attraverso strumenti di tecnologia e di intelligenza artificiale. L'mRNA, cioè lo strumento che ha permesso il vaccino, è una tecnologia che applicata al tumore o all'HIV può arrivare a risolvere definitivamente il problema di alcuni settori e di alcune forme tumorali.

Negli ultimi vent'anni le aziende italiane - quelle che venivano definite piccole e medie imprese e che dovevano fallire secondo i grandi esperti economici - sono cresciute. Tali aziende sono cresciute e hanno fatto acquisizioni. Guardatevi i *report* di Farmindustria. È una realtà che occupa 70.000 persone

Ma per ridurre le liste d'attesa devi innanzitutto chiarire a te stesso qual è la riorganizzazione che immagini, quanta tecnologia vuoi mettere e quali investimenti vuoi fare in prospettiva. Da qui a vent'anni, infatti, vivremo tutti più a lungo, o almeno ce lo auguriamo (l'età media sicuramente crescerà) e cambierà totalmente il modello di organizzazione della sanità. Prima la collega Gelmini raccontava il cambiamento fatto da Tony Blair nella sanità inglese. Proprio qualche giorno fa Tony Blair presentava per il Governo Starmer, il nuovo governo laburista del Regno Unito, un modello in cui l'intelligenza artificiale porta nella prevenzione a migliorare di gran lunga

ma è anche, con il cuore in mano, un invito a questo Senato: quando si parla di sanità, non si parla di un problema come gli altri, perché chi ha un problema sanitario da noi si aspetta risposte all'altezza della propria sfida. Se tu hai un tumore o una diagnosi di Parkinson, non vuoi che il Parlamento si metta a discutere per prendere tre *like* o tre voti in più; ti aspetti che quel Parlamento sia all'altezza dei sogni e delle aspettative degli italiani. Io penso che come organizzazione, come capitale umano, come ricerca, come dimensione industriale e persino come ecosistema legato alla finanza e al *venture capital* legato alla sanità, noi possiamo fare molto di più, però bisogna avere un Parlamento della Repubblica che su questi temi gioca con parole da adulti e non con l'atteggiamento di reciproci *spot* che la maggioranza ha imposto, scegliendo di fare un decreto-legge nella settimana elettorale. Che ci fossero le liste d'attesa, cara Presidente Meloni, ve ne siete accorti soltanto a dieci giorni dalle elezioni? E siccome poi non siete riusciti a trovare un accordo, ci avete fatto passare le giornate in attesa di trovare il vostro accordo sul benedetto articolo 2: siete davvero convinti che quello non fosse uno *spot*? Allora, giocate da adulti e troverete la nostra collaborazione e la nostra sfida. Se continuate con gli *slogan*, state prendendo in giro non noi, perché potete farlo,

Scherzavo, perché non stava disturbando così tanto. Forse era Lotito che disturbava più di Renzi.

Ad esempio, non ho sentito una parola in questa discussione sul ruolo dei medici di famiglia. Forse sono

però un fatto preliminare che va affrontato: ogni Regione ha il suo sistema, il suo modo di operare, *ergo* bisogna affrontare quel tipo di tema.

probabilmente sono meglio pagati, probabilmente hanno un trattamento diverso. E noi pensiamo di risolvere il problema delle liste d'attesa aumentando gli straordinari, facendo lavorare il sabato e la domenica. A me pare un'impostazione sbagliata: è un'opinione, ma posso non essere d'accordo su una cosa che - a mio avviso - non risolverà niente da questo punto di vista? Si dice che, per fare questo, ci vogliono le risorse.

anche perché i soldi sono dei cittadini e delle cittadine italiani, di quelli che pagano le tasse. Quindi, lo Stato deve spendere meglio da questo punto di vista. Però che senso ha? Se uno guarda le classifiche, il ragionamento è sul rapporto tra PIL e spesa sanitaria;

il tema e cerchiamo ognuno di dare un contributo che va in una certa direzione, oppure pensiamo che basti fare un decreto propagandistico - come ho detto - perché è così; addirittura si affermava che si poteva abbattere il blocco della spesa sanitaria. Questo era scritto ed è stato dichiarato, ma non c'è. Infine,

che - l'ho detto anche ieri - un emendamento a mia prima firma e del mio Gruppo era uguale all'emendamento presentato dalla Lega; se avessimo votato, in questo caso sarebbe andato sotto il Governo.

Innanzitutto, bisogna evidenziare che questo decreto-legge ha un merito evidente ed immediato: quello di aver messo al centro dell'attenzione parlamentare il tema delle liste di attesa. Il decreto-legge entra puntualmente nel merito dei problemi della sanità, che causano le liste d'attesa, proponendo delle soluzioni, alcune immediatamente vigenti, altre che necessitano di disposizioni applicative, altre che vengono anticipate e che faranno parte del complesso di norme che formeranno il pacchetto sanità in occasione della legge di bilancio. È evidente a tutti che la stagione di un sistema complesso come il Servizio sanitario nazionale, assieme a ventuno sistemi regionali, dovrà passare attraverso la manovra per il 2025 e gli anni successivi, perché manifesto a chiunque che il Sistema sanitario pubblico necessita di risorse economiche per essere migliorato. Anche la riscrittura dell'articolo 2, durante l'esame della Commissione affari sociali, ha dimostrato quanto la dinamica Regioni-Stato sia sempre presente. Le Regioni custodiscono gelosamente le proprie competenze, la sanità necessita di migliori condizioni stipendiali per chi vi lavora, spesso con enorme spirito di dedizione e sacrificio, anche per evitare l'esodo verso l'estero delle figure più qualificate. Ecco che la manovra, che detassa gli straordinari dagli operatori sanitari, certamente va già nella stima della maggiore disponibilità oraria dei medici e infermieri. Ma il sistema sanitario necessita anche di un complesso intervento di organizzazione degli spazi e delle strutture dedicate alla salute dei cittadini. Al contempo, come abbiamo visto, in alcune Regioni il modello organizzativo del privato convenzionato funziona e, soprattutto, rappresenta un forte stimolo a migliorare quello delle strutture pubbliche. Certamente il tema che rimane è mettere in campo le verifiche più opportune sulle liste d'attesa, anche su segnalazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. Altro passo in avanti è l'adozione di linee guida omogenee in tutta Italia sui sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione; così come si prevede che vi siano agende dedicate per le prestazioni dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali In tal senso, non si potranno chiudere o sospendere le attività di prenotazione che riguardano i livelli essenziali di assistenza e si pongono le basi per dare garanzia all'erogazione delle prestazioni utilizzando l'attività professionale intramuraria, ma anche il privato accreditato con le tariffe nazionali vigenti. Bene, come detto, l'imposta sostitutiva del 15 per cento sugli straordinari: è un incentivo concreto e fa sì che ci si trattenga di più in ospedale senza dover perdere buona parte del premio della propria abnegazione. Sappiamo benissimo che l'aliquota marginale, cioè quella più alta, sostanzialmente dimezza il guadagno dello straordinario e quello non è certamente un incentivo a restare in corsia. Come diceva il presidente Berlusconi, c'è un momento dell'anno in cui si smette di lavorare per lo Stato e si comincia a lavorare per sé stessi. Ora si anticipa quel momento, almeno per il personale sanitario. Inoltre, poter lavorare anche il sabato e la domenica significa utilizzare non solo la forza lavoro, ma anche gli spazi e le macchine per la diagnosi in modo più completo. Si mettono quindi a fattore comune una pluralità di esigenze. Spesso le strutture e le macchine pubbliche vengano utilizzate per l'attività libero-professionale. Prevedere un rapporto più equilibrato tra le esigenze dei professionisti, il loro reddito e lo smaltimento delle attività istituzionali è un altro passo in avanti. Si affronta quindi il tema della contrattazione integrativa da parte delle Regioni e delle Province autonome, che potranno valorizzare la professionalità di chi opera in ambito sanitario. Sono previste deroghe per potersi avvalere degli specialisti ambulatoriali già in servizio a tempo indeterminato ed è previsto l'aumento delle paghe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico. Importante - a nostro avviso - è anche la possibilità per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario di reclutare personale sanitario con contratto di lavoro autonomo. Viene poi affrontato il tema dei temi, quello della appropriatezza prescrittiva, posto che alcuni studi e *report* ritengono che le prescrizioni non appropriate siano addirittura una ogni tre. Attribuire alle prescrizioni una classe di priorità certamente può contribuire a smaltire le liste. Perfino il maggiore coinvolgimento dei cittadini sarà l'occasione per segnalare i disservizi delle strutture della sanità nella gestione delle liste. Un più puntuale coinvolgimento dei privati accreditati è un'altra via che va certamente percorsa ed è un altro modo per liberare le strutture ospedaliere che forniscono servizi simili. Abbiamo inoltre apprezzato l'ascolto che la Commissione presieduta dal presidente Francesco Zaffini ha voluto dare agli esperti, alle associazioni dei lavoratori e dei pazienti, che hanno portato ciascuno la propria esperienza utile a completare il quadro normativo per affrontare in modo serio e non demagogico un problema che ogni giorno tocca la pelle dei cittadini. Valutiamo inoltre positivamente l'accoglimento di diversi articoli proposti da Forza Italia, che ci auguriamo ora trovino attuazione nei prossimi provvedimenti. Ci rendiamo infatti perfettamente conto che alcune misure di questo decreto sono immediatamente operative, che altre invece necessitano delle disposizioni attuative e che altre ancora dovranno essere aggiunte, come peraltro ha già anticipato il ministro Schillaci. Valutiamo il lavoro fatto finora certamente molto apprezzabile, in quanto segna un fondamentale cambio di passo verso una sanità più efficiente e più equa su tutto il territorio italiano. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

devo confessarvi che ieri durante il dibattito mi sono sentito a disagio, perché ho ascoltato da questa maggioranza che il Sistema sanitario nazionale, tutto sommato, è in buona salute, dato che siamo uno dei Paesi più longevi al mondo e che quello che è stato fatto è il meglio di quello che si poteva fare; anzi, è stato fatto qualcosa che nessuno mai aveva fatto: il finanziamento maggiore in termini assoluti. Si è dimenticato di dire, però, che è solo in rapporto al PIL che a livello internazionale si comparano i sistemi e che proprio in rapporto al PIL non è prevista alcuna crescita di spesa, ma è previsto un costante e lento sottofinanziamento. A rafforzare, però, questa visione positiva del Sistema sanitario nazionale, la senatrice Musolino ha citato un sondaggio dell'istituto Piepoli che titolava: decreto liste d'attesa promosso dall'86 per cento degli italiani. Peccato però che la senatrice si è fermata al titolo senza approfondire, senza leggere le risposte che hanno dato gli italiani. Ebbene, il 41 per cento del campione ritiene che una delle tre misure più efficaci sia l'attivazione di un organismo di verifica e controllo presso le ASL per garantire il corretto funzionamento della gestione delle liste d'attesa con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria. Proprio su questo punto, però, il ministro Schillaci e il Governo hanno dovuto fare marcia indietro. Il testo che approverete non ha più questo indirizzo, che è uno dei principali motivi per i quali l'opinione pubblica apprezzava questo decreto-legge.

Più scendiamo nel dettaglio e più emerge una realtà diversa da quella che ci è stata rappresentata qui agiograficamente, beatificando il ministro Schillaci. Quale sarà il terzo motivo che spinge l'opinione pubblica a essere favorevole verso il decreto-legge in esame? È semplice: la possibilità di fare gli esami diagnostici nei *weekend.* Tutti siamo felici di ciò, ma per questa estensione di lavoro non sono previste nuove assunzioni: gli stessi operatori sanitari, tecnici di laboratorio, infermieri e operatori sociosanitari, gli stessi che hanno l'età media più alta d'Europa lavoreranno anche il sabato e la domenica. Ciò rende l'applicazione pratica della misura molto limitata: è uno spot pubblicitario senza personale e senza risorse aggiuntive. saputo che tre delle misure ritenute più efficaci (tre su tre in realtà) non si possono realizzare e certamente non si realizzeranno, quale avrebbe potuto essere il risultato del nuovo sondaggio? Come si sentiranno oggi gli italiani? Le lunghe liste d'attesa per visite specialistiche ed esami medici - come sappiamo - hanno causato e causano gravi ritardi nell'accesso alle cure: due milioni di persone hanno rinunciato a qualsiasi forma di cura. Purtroppo, l'aver snaturato l'indirizzo e le indicazioni contenute nel decreto-legge e l'aver messo la museruola al ministro Schillaci per tenere buono l'alleato Salvini non promettono nulla di buono per gli italiani, che hanno rinunciato alle cure per lunghi tempi di attesa. Siamo delusi del fatto che le soluzioni da noi proposte non siano state prese in considerazione e che la problematica della sanità venga affrontata in modo così superficiale. Questa è un'opportunità persa per fare qualcosa di utile al Paese, invece di usare i decreti-legge per fini propagandistici. In sintesi, se non ci fosse stata questa situazione ostativa, avremmo potuto lavorare in Commissione per migliorare il provvedimento; invece siamo stati costretti ad aspettare il parere delle Regioni, che hanno ribadito la gestione regionale della sanità e il ruolo dello Stato nell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Il Governo ha dovuto cedere alle Regioni nella stesura di una parte fondamentale del decreto-legge, ridimensionando il controllo da parte del Ministro della salute sulle liste d'attesa, evitando così l'invasione di campo. Questa non è già una rappresentazione plastica del conflitto Stato-Regioni che la scelta di un'autonomia regionale differenziata, imposta dalla Lega a questa maggioranza, acuirà ulteriormente? In prospettiva è evidente che la scelta di concedere maggiore autonomia alle Regioni potrà esacerbare ulteriormente il conflitto Stato-Regioni, indebolendo l'azione dello stesso Esecutivo e, comunque, alimentando ulteriori conflitti tra le Regioni e lo Stato centrale, con possibili ripercussioni sulla coesione e l'unità del Paese. Un Consiglio dei ministri che licenzia un testo, poi sbugiardato dai Presidenti della Regione, non perde di credibilità? Eppure il presidente Rocca ha dimostrato di voler affrontare il problema reale delle liste d'attesa, che è il potenziamento delle risorse del personale sanitario e la gestione del Fondo sanitario nazionale. Questo ci suggerisce che sta cercando una soluzione concreta e non sta solo facendo dichiarazioni vuote. Il presidente Rocca, appartenente a Fratelli d'Italia e non certo una persona di sinistra, in Commissione ha chiesto un punto di caduta per affrontare il vero problema delle liste d'attesa, che è quello del potenziamento delle risorse del personale sanitario e della gestione della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Dove lo dice? Dove si afferma questo? Lo si afferma nel documento della Conferenza Stato-Regioni, dove si scrive nero su bianco che, per avere un'efficace attuazione delle misure di contenimento dei tempi di attesa, è necessario disporre di congrue risorse economico finanziarie aggiuntive e di adeguate risorse umane. Ripeto: lo dicono le Regioni e noi, come Gruppo, abbiamo proposto emendamenti esattamente in linea con queste affermazioni delle Regioni, e cioè l'incremento del Fondo sanitario nazionale, l'istituzione di un fondo per un piano straordinario di assunzioni e di personale medico. Presidente, per il suo tramite, dica alla presidente Meloni che la diagnosi è corretta, ma la terapia è sbagliata. Serve un Piano Marshall di assunzioni per abbattere le liste d'attesa. Basta *spot* propagandistici sulla pelle delle persone. Basta bugie, *slogan*. Manca tutto quello che vi abbiamo detto. Questo provvedimento è un piatto vuoto. quale credibilità può avere un Governo che - da un lato - sventola la bandiera delle autonomie differenziate, accentuando la disuguaglianza tra le Regioni e - dall'altro lato - propone un provvedimento che nella formulazione originaria - ribadisco - così come uscito dal Consiglio dei ministri, avrebbe realmente ed efficacemente implementato un sistema di governo delle liste d'attesa di livello centrale, superando le attuali frammentarietà dei diversi sistemi regionali, in una cornice di effettività e di efficienza dell'offerta assistenziale e nella tempestività dell'accesso ai LEA, materia indiscutibilmente di competenza esclusiva di cui all'articolo 117, comma 2, Il Governo, ostaggio della Lega, ha presentato un emendamento abrogativo dell'articolo 2, nucleo essenziale delle garanzie minime che avrebbero assicurato la tutela del diritto alla salute a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. Il Ministro della salute ha tentato invano di dare effettiva cogenza a norme che erano già declamate nel piano nazionale di gestione delle liste d'attesa, che ora conserva un potere d'accesso presso le ASL, limitato limitato alla verifica di efficienza e appropriatezza dei LEA, mentre è nata una figura nuova, il responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria, che che in sostanza è un vero e proprio parafulmine dell'assessore o dei presidenti della Regione, che provvederà a valutare i conseguenti interventi. Insomma, un pasticcio: se c'era qualcosa da peggiorare, ci siete riusciti. Quindi niente più visite ispettive, come voleva il Ministro; niente più segnalazioni dei cittadini o associazioni di categorie, come voleva anche il Ministro, come volevamo noi e come abbiamo proposto nei nostri emendamenti. Niente più segnalazioni di irregolarità, niente più sanzioni o premi per i responsabili regionali e neanche più la possibilità di revocare l'incarico, solo in caso di mancata nomina del parafulmine RUAS o in caso di ripetute inadempienze. Non si capisce poi quante siano le ripetute inadempienze. Il Ministro, attraverso l'organismo di verifica e controllo, potrà agire con poteri sostitutivi.

abbiamo bisogno di fondi effettivi, mentre assistiamo ad una forma di sfruttamento dei professionisti, ai quali vengono negate le progressioni di carriera; non li valorizziamo economicamente e professionalmente. In questo decreto cosa volevamo fare, senza aumentare il personale sanitario e senza invertire la rotta? Allo stesso personale sanitario, stremato, demotivato e in fuga, chiediamo di fare gli straordinari

…se acquistare 22 cacciabombardieri, per una spesa di 7 miliardi, invece di potenziare il personale sanitario. *(Applausi)*. Per i cacciabombardieri i soldi li trovate, per il personale sanitario no. Io vi regalo questo giocattolo: giocate con il cacciabombardiere giocattolo e non con la pelle delle persone!

quanto il problema delle liste d'attesa si sia cristallizzato nel tempo, perché tutti noi ne siamo consapevoli. Vorrei però farvi riflettere sul fatto che non ci può essere un unico fattore risolutivo, data la molteplicità causale che le ha generate, ma più verosimilmente - come ho avuto già modo di proporre e non mi stancherò mai di rifarlo - una pluralità di fattori combinati, supportati da interventi legislativi ordinamentali e settoriali, con nuove regole di ingaggio degli erogatori e dei prescrittori. Il decreto-legge n. 73, in conversione, è uno di questi, pur nella consapevolezza della sua relatività. Ma facciamo un passo indietro. Molta dell'utenza che è in lista d'attesa è in età avanzata. Non vorrei entrare in un pregiudizio ageistico, ma l'età avanzata può voler dire diventare ipocondriaci e può avere a che fare, talvolta, con una perdita di memoria. Nel secondo caso, ci troviamo di fronte a un possibile utente che, a distanza di mesi, ha dimenticato il suo appuntamento. E il *remind* è una buona soluzione, ancorché sanzionata in caso di mancata presentazione. Se il pagamento del *ticket* può portare delle risorse nelle casse del sistema, è lo scorrere della graduatoria, secondo le nuove misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, con una graduatoria dedicata alle indifferibili ed urgenti, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi e da cui pescare per tutti gli *slot* che si vanno liberando, che potrebbe contribuire fattivamente alla normalizzazione dei tempi di attesa urgenti e delle relative liste. Nel primo caso ci troviamo di fronte a una situazione tale per cui, soprattutto se di paziente cronico ed anziano, che, avendo tempo libero e ansia di longevità in salute, quindi di stare bene, nei suoi argomenti di conversazione prevalenti tra coetanei vi è proprio il parlare di sanità, concausa di iperprescrizione. Banalmente esemplificando, se il mio vicino ha fatto una risonanza magnetica alla spalla e me ne parla bene, stante che anch'io ho dei piccoli dolorini ogni tanto alla spalla, può venirmi in mente di fare la stessa cosa: vado dal mio medico e chiedo di prescrivermela, senza averne effettiva necessità. Il medico, per effetto di quella che viene definita medicina difensiva, anziché provare a fare anamnesi, è portato a fare la ricetta. Ora, non nascondiamoci dietro un dito: molte volte la ricetta viene predisposta dall'infermiere. E il medico, stressato dagli innumerevoli adempimenti burocratico- amministrativi, procede di conseguenza. Ecco, qui entriamo nel cuore del capitolo che ho cercato più volte di rappresentare: se con le risorse del PNRR pensassimo di dotare in comodato d'uso i medici di medicina generale di strumenti analitico-diagnostici di primo intervento, coadiuvati, in caso di dubbio, dal *second opinion supporting* specialistico, e si andasse a ridurre il numero degli assistiti per ciascun medico, facendo leva su misure di reclutamento flessibile e immediato incremento quanti-qualitativo delle attività in studio e a domicilio, nel frangente del potenziamento strutturato dei 10.000 medici che mancano all'appello - così come previsto nei nostri disegni di legge nn. e con i modelli prototipali settorialmente indicati per le patologie oculari cronico-degenerative nel n. 483, e per le patologie reumatologiche ad elevato carico invalidante nel disegno di legge n. 946, oltre a quanto apprezzabilmente contenuto nel disegno di legge governativo - andremmo ad approcciare organicamente e definitivamente il problema nella sua complessità, emergenza-urgenza compresa, in una dinamica integrata fra sistema ospedaliero ed extraospedaliero, in parte contribuendo anche al disintasamento dei pronto soccorso. La strategia di sviluppo evolutivo del nostro Servizio sanitario nazionale dovrebbe significare che una parte importante dei bisogni espressi viene presa in carico fuori dall'ospedale e dalle liste d'attesa, superando la deresponsabilizzazione che, sommata a sanità divulgata da fonti talvolta non altamente qualificate, contribuisce al cosiddetto consumismo estremo in sanità. La controprova è che il vero tema è la corretta e oculata finalizzazione delle risorse disponibili, con effetto moltiplicatore e generatore di valore, attraverso la tracciabilità, la valutazione e il controllo degli impieghi e degli esiti, in ossequio al generale principio "dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio", superando la dicotomia controllore-controllato. Da qui la necessità di una forte *governance* pubblica nella prevenzione, programmazione e acquisto delle prestazioni sanitarie di tutti gli erogatori in rete, secondo flussi informativi parlanti, vale a dire dati e informazioni opportunamente calibrati, contenenti gli elementi essenziali per l'analisi, la valutazione del controllo delle *performance*; incentivando le pratiche virtuose e remunerando adeguatamente prevenzione e appropriatezza, certi che si possa realizzare, recependo le cinque regole fondamentali indicate nell'articolo 2 del nostro disegno di legge n. 1153. Ed è per tutto quanto detto e nonostante tutto che la nostra è una dichiarazione di voto favorevole. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, si dice che la strada dell'inferno sia lastricata di buone intenzioni. Il modo di dire, molto caro alla famiglia dei Padri salesiani, si attaglia davvero molto bene al decreto-legge che ci apprestiamo a votare. È l'ennesimo decreto (siamo al numero settanta), ed è il primo sulla sanità. norme che dovrebbero dare risposta a un problema drammatico come quello delle liste d'attesa, causa di un grande disagio quando non di veri e propri calvari per i cittadini: 10 milioni di prestazioni inevase e 4 milioni di persone che rinunciano a curarsi. Il Governo ha annunciato il provvedimento a gennaio e lo ha licenziato il 7 giugno in pompa magna, presentandolo come una rivoluzione: non poteva attendere che si concludesse la campagna elettorale. A oltre un mese di distanza, dopo aver assistito a un vero e proprio gioco di ricatti e sgambetti politici tutti dentro la maggioranza, reduci da giorni inconcludenti per l'incapacità del Governo di fare i passi necessari per arrivare almeno a concludere l'*iter* parlamentare, siamo chiamati oggi al voto finale. Voglio spiegare bene perché noi bocciamo questo decreto, sbagliato per il metodo, ma soprattutto per il suo contenuto. Siamo di fronte a qualcosa che sembra più una presa in giro che un tentativo di risposta; si badi bene, una presa in giro non nei confronti dell'opposizione, che è stata disponibile sempre a discutere soluzioni. Si è vista la vostra attenzione dal metodo con cui avete bocciato tutti tutti gli emendamenti, salvo renderne una grande parte assolutamente improponibili, quindi neanche degni di essere discussi. Continuate così, non ascoltate. Non potrebbe che essere così: l'opposizione c'è sempre, quando c'è in gioco la salute dei cittadini. Questo decreto-legge è una presa in giro degli italiani, dei medici del Servizio sanitario nazionale, di tutti i lavoratori della sanità e di quanti credono in quello che fanno quando si prendono cura delle persone e dei loro problemi. Si è consumato uno scontro duro tra il Governo e le Regioni, che, ci piaccia o meno, hanno in mano l'organizzazione e il funzionamento della sanità; tale scontro lascia esterrefatti, perché si è prodotto dentro una maggioranza politica che approva, contro tutto e contro tutti, una riforma dell'autonomia che, una volta a regime, malauguratamente, negherebbe ai cittadini un uguale diritto alla salute. Dall'altra parte,

ossia risorse finanziarie e di personale. Un minimo di serietà! Si resta ancora più esterrefatti per il livello di improvvisazione con cui si è agito. Ma come fa un Ministro, anche oggi assente da quest'Aula - e parliamo del primo decreto-legge sulla sanità del ministro Schillaci,

Ebbene, il risultato è stato ben spiegato: è un testacoda e una soluzione pasticciata, che darà origine a confusioni di ruolo e a contenziosi. Niente di buono per le liste d'attesa, ma soprattutto per i cittadini in attesa. E veniamo al resto: il provvedimento si concentra solo sui sintomi e non sulle cause delle liste d'attesa, che richiedono dalla politica una decisione vera su spesa e personale. Pensate davvero che senza soldi, con una progressiva riduzione delle risorse già insufficienti (ve l'ha detto anche ieri la Corte dei conti) e chiedendo al personale di fare di più, sempre di più, senza mettere mano al tetto di spesa sul personale, istituito nel 2005 dal Governo Berlusconi, si possa andare da qualche parte? Lo credete davvero? Io penso che voi sappiate che non è vero: non si va da nessuna parte. Il capolavoro lo riscontriamo all'articolo 7, che prevede la defiscalizzazione dei compensi per le prestazioni aggiuntive, una misura finanziata interamente con i fondi del Servizio sanitario nazionale: sembra il gioco delle tre carte. Sia chiaro: riconoscere il valore del lavoro che svolge il personale del Servizio sanitario e iniziare ad aumentare le remunerazioni è un obiettivo che condividiamo assolutamente e che potrebbe costituire davvero un elemento strutturale per rafforzare il Servizio sanitario ma dal provvedimento non traspaiono questi obiettivi. La scelta è semplicemente quella di dare un segnale (non dimentichiamo che il decreto è pre-elettorale), estendendo anche a loro l'abbattimento del prelievo fiscale già delineato dal Governo in altri ambiti. Tale incentivo è stato accolto positivamente dai rappresentanti della categoria, stremati dalle difficoltà in cui versano, ma che presenta molte criticità: è poco efficace, posto che sui professionisti gravano pesantissime condizioni di lavoro. Guardate che la gran parte dei lavoratori della sanità sono donne, a cui chiedete, oltre che di fare

contribuisce a destrutturare ulteriormente il sistema fiscale. Andiamo pure avanti così, ma vorrei sapere la sanità chi pensiamo che la pagherà. Lo stato attuale della sanità pubblica richiede scelte in grado di avviare con determinazione il superamento degli ostacoli che rendono difficile, in molte realtà, rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone, ricostituire la fiducia dei cittadini e restituire anche un minimo di credibilità. È una situazione nella quale i medici, gli operatori sanitari e i lavoratori, che sono veramente allo stremo delle forze, anche psicologicamente, si sentono presi in giro. Devono tornare a sentire che la loro è una missione. Questo decreto-legge riduce tutto a un fatto contingente, mentre le debolezze della sanità pubblica non sono niente affatto transitorie e richiedono interventi di sistema. L'unico intervento strutturale, contenuto nel decreto-legge, com'è stato detto poco fa, riguarda l'istituzione di una piattaforma nazionale, volta a superare questi limiti del sistema di monitoraggio. È uno strumento condivisibile, la cui realizzazione richiede però non solo tempi molto lunghi, ma una capacità di dialogo con le Regioni che mi sembra abbia mostrato qualche falla, visto che sono le Regioni che si sono contrapposte al decreto-legge e hanno impedito per quindici giorni che si andasse avanti. Visto che sono qui, ne approfitto per rivolgervi un invito, anche dopo avervi ascoltato questa mattina e ieri. Vi ascolto sempre con rispetto e attenzione, però ve lo voglio dire sinceramente: fatela finita con la lagna che è tutta colpa di chi c'era prima. *(Applausi)*. che voi vorreste fare qualcosa di buono, ma quelli che c'erano prima vi hanno lasciato tutto rotto e guasto. Guardate, è un giochino tale per cui prima la gente non vi ascolterà neanche più. Fatela finita per due ragioni: prima di tutto, perché c'eravate voi, tutti insieme, nel Governo Berlusconi che ha messo il tetto sul personale

Penso che dopo due anni si abbia il dovere di governare e di dimostrare a chi vi ha eletto e anche a chi non vi ha eletto *(Applausi)*. Lasciate che vi dica che impressiona vedere tanta improvvisazione e tanto cinismo. In conclusione, noi abbiamo potuto studiarlo questo decreto-legge e oggi siamo nelle condizioni di denunciarne l'inefficienza e l'inefficacia.

anch'essi un po' vittime del lavoro che la Commissione ha dovuto svolgere per portare avanti questo decreto-legge. Mi lasci ringraziare il relatore, i colleghi, ovviamente di entrambe le cosiddette parti, quindi maggioranza e opposizione,

Presidente, il tema è annoso, la *vexata quaestio* delle liste d'attesa, uno dei tanti temi che appesantiscono il nostro Sistema sanitario nazionale, anche se non è il solo, e che viene ovviamente da molto lontano. Ricordo ai colleghi una una curiosità storica: l'allora presidente Formigoni, molti anni fa, inventò la sanità privata convenzionata per assorbire le liste d'attesa, che

Le liste d'attesa, però, sono lì e sono anche aumentate rispetto ad allora, quindi il problema non è risolto, eppure il Servizio sanitario nazionale è profondamente cambiato. Cito questo episodio non per almanacco, ma perché sul tema delle liste d'attesa si sono fatte anche riforme importanti del Sistema sanitario nazionale, non riuscendo a risolverlo. Questo

l'ultima delle quali - la più recente, probabilmente - è l'inappropriatezza prescrittiva e terapeutica. Cito solo un dato, che abbiamo appreso dalle audizioni:

È genericamente il Sud quello che sta indietro, ma abbiamo anche qualche sorpresa in Regioni del Nord, come quella del presidente Fedriga, per esempio, per dirne una solo a caso. inappropriatezza, non equa distribuzione dei LEA e del nostro sistema di prestazioni e di erogazione delle prestazioni.

di prestazioni erogate attraverso i professionisti, che non ci sono: non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, non ci sono gli operatori sociosanitari e non ci sono i tecnici sanitari. Tutte le professioni sono paradossalmente mancanti di professionisti. È facile dire, collega Zampa, Zampa, di farla finita, però è anche difficile gestire un sistema in cui certamente sarebbe opportuno assumere, in cui la capacità assunzionale delle Regioni è stata aumentata con diversi provvedimenti anche durante il Covid, ma in cui le Regioni non sono riuscite ad assumere, perché non ci sono le figure utili a rispondere ai concorsi che vengono banditi.

Era un'ipotesi, ma questo Governo non lo ha fatto, come ieri ha detto molto bene il collega Zullo, il relatore del provvedimento. Questo Governo ha deciso intanto di agire in via d'urgenza. Questo è il motivo del decreto-legge:

ottenendo anche risultati importanti. Vi posso citare l'Umbria, che in questo momento ha assorbito bene (diciamo il meglio possibile) le liste d'attesa, tanto da essere la terza

in parallelo - non lo ha promesso, ma lo ha approvato in parallelo - un disegno di legge di iniziativa governativa che arriverà in Parlamento i primi di settembre, appena riprenderemo l'attività. Il primo è un provvedimento d'urgenza, soprattutto di natura organizzativa, ed è evidente che su un provvedimento del genere non si non si possono mettere risorse assolutamente rilevanti, perché attinge alla programmazione reale, esistente e di quel momento. Nel disegno di legge di iniziativa governativa potremo stanziare risorse aggiuntive, perché andremo auspicabilmente ad attingere alle programmazioni del 2025. Tuttavia, colleghi, non è vero che in questo provvedimento non c'è danaro,

stati attinti dai fondi del Ministero per il compenso del lavoro fuori orario dei professionisti. Certo, collega Magni, che noi spingiamo gli attuali professionisti a darci più disponibilità: è necessario farlo, non avendo a disposizione

reddito del professionista, consente di avere un grande beneficio. Altri 624 milioni di euro sono stati messi come fondi del PNRR e sono andati per l'assorbimento di liste d'attesa, ma potevano andare in qualunque altra fonte di spesa del Servizio sanitario nazionale.

Personalmente, condivido quello che ha detto il collega Mazzella: anche io avrei preferito il testo uscito e votato da tutto il Consiglio dei ministri. È evidente però che, in una logica di sana e corretta collaborazione tra Istituzioni dello Stato, lo sforzo che è stato compiuto per trovare l'accordo in Conferenza Stato-Regioni è auspicabile.

ai colleghi di smetterla di dividerci sui temi attinenti alla salute, perché questo procura un danno enorme al nostro Servizio sanitario, alla dignità dei nostri professionisti e alla correttezza dell'informazione che diamo

Fiori, scomparso martedì all'età di ottantasei anni. Publio Fiori è un uomo delle Istituzioni, ha fatto per sette legislature il parlamentare, è stato vice presidente della Camera e Ministro dei trasporti nel primo Governo Berlusconi. Ho avuto l'onore di conoscerlo quando già era una persona nota e importante. Peraltro nel 1977 era stato attinto da colpi di arma da fuoco delle Brigate rosse, che lo avevano in qualche modo cercato di intimorire (o, forse, di uccidere). È notorio che chi lo soccorse per primo, credendo che stesse per morire, gli disse «ricordati che Dio è buono» e lui rispose «sì, lo so, Dio è buono, ma chiama l'ambulanza». Doveva assolutamente dire così. Era democristiano. Io l'ho conosciuto nel 1993 1993 quando Fini si candidò a Roma come sindaco e lui lo appoggiò senza essere candidato. Fu poi tra i costruttori di Alleanza nazionale, perché credeva in un Parlamento in cui destra, sinistra e centro potessero confrontarsi democraticamente. È sempre stata la sua ambizione. L'ho visto anche pochissimo tempo fa, quando stava lavorando a mettere insieme un Centro democratico che potesse servire a far trovare al Parlamento occasioni di confronto sempre più sincere e democratiche. La nostra amicizia è durata fino alla fine. La sua capacità di ascolto e di fare politica, soprattutto di ascolto verso chi non la pensava come lui, è rimasta proverbiale. Vorrei ricordarlo a tutti voi, perché ci lascia un amico, un esponente importante della politica, e rinnovo anche da parte di tutti voi il nostro cordoglio ai suoi familiari e gli mando un affettuoso saluto, perché sono certo che in questo momento sta guardando anche alla nostra Aula. Grazie, Publio.

Grazie,